Avverto che, come già annunciato all'Assemblea, immediatamente dopo il voto sulla questione pregiudiziale si passerà alla votazione del documento IV-*bis*, n. 2 della Giunta delle elezioni

Siamo, in realtà, perfino di fronte ad un nome che è tralaticio, come l'editto del pretore nel diritto romano. Non a caso c'è un «mille proroghe» ogni anno. È un decreto che risponde all'esigenza di compattare un insieme di questioni, anche assai diverse, ma tutte accomunate dal profilo di avere un elemento di temporalità come connotazione qualificante. Certo - lo comprendo -, può darsi che non sia una buona prassi, ma di sicuro è, appunto, una prassi. Può darsi che sia una prassi che denota anche una disfunzione di sistema - è possibile -, ma

(sul quale apprezzo l'indirizzo stamattina manifestato dalla Presidenza), che per altro non sono oggetto della nostra valutazione in questo momento. Si censura il fatto che, nell'ambito di questo complessivo disegno di proroghe, ci siano singole norme che non sono proroghe, o che si proroghino termini già scaduti. Questi, in particolare, sono due profili oggi evidenziati mi pare dal collega Pastore. Sul primo punto c'è però da dire che nessun decreto‑legge, e nessun atto in generale, si ritiene possibile che venga in ogni sua parola, in ogni suo rigo, segnato dalla stretta aderenza a quella che è la connotazione generale del testo. Certamente in un decreto‑legge non ogni parola ha il requisito della necessità e dell'urgenza; allo stesso modo, in questo decreto non ogni rigo ha tecnicamente a che fare con il superamento di un termine, la decorrenza di una data. L'importante è che, nell'insieme e in maniera

delle proroghe di termini già scaduti e, quindi, come tali, tecnicamente non sono prorogabili. In un caso di questo genere, in realtà, la

una disciplina normativa nuova. Quindi, in realtà, in questo caso ci troviamo di fronte ad una di quelle ipotesi in cui, nell'ambito di un testo complessivamente volto alle proroghe, abbiamo un qualcosa che proroga, da

in specie un problema sui direttori degli istituti del CNR che vengono prorogati fino ad una certa data sospendendosi, contestualmente, le procedure concorsuali. Non mi sembrano decisive le considerazioni che siano termini non previsti da previsione legislativa: è un rilievo esclusivamente formale che certamente non assume un peso significativo.

oggetto fa esplicito riferimento al riordino del CNR e, allora, il senso della sospensione delle procedure si trova guardando, appunto, alla prospettiva del riordino, rispetto al quale, ovviamente, non si può parlare (ho sentito un collega che oggi poneva questo argomento) di un diritto di qualcuno a sostituire i direttori. Non c'è ovviamente nessun diritto da parte di chicchessia; ci può essere una legittima aspettativa nell'ambito di un quadro di regole dato, ma non c'è alcun diritto tutelabile nei confronti di un quadro che venga ad essere modificato.

ma di una misura che assume il dato temporalmente definito come fondamento per l'adozione di una disciplina normativa,

nonché dei signori Marco Preioni, Daniela Bianchini, Fausto De Santis, Alfonso Papa, Monica Tarchi, Settembrino Nebbioso e Alberto Uva, ciascuno *in parte qua*, per i reati di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio)». Nella seduta antimeridiana si è esaurita la fase della discussione e delle dichiarazioni di voto. Ai sensi dell'articolo 135*-bis*, comma 8*-bis*, del Regolamento, il risultato delle votazioni che ora effettueremo non sarà immediatamente proclamato in quanto i senatori che non abbiano potuto partecipare a questo voto elettronico, né a quelli successivi, potranno comunicare il proprio voto ai senatori segretari

Passiamo alla votazione

Dichiaro chiusa la votazione.

proprio voto ai senatori segretari. Ricordo nuovamente che i senatori che non abbiano potuto partecipare alle votazioni elettroniche potranno comunicare i propri voti ai senatori segretari che ne prenderanno nota in appositi verbali; la procedura rimarrà aperta sino alle ore 19,30.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà. Signor Presidente, mi soffermerò brevemente su un solo punto di questo complesso provvedimento, molto composito. Il punto è quello di cui ha già parlato il senatore Possa questa mattina presentando una pregiudiziale; si tratta dell'articolo 1, dove si dice: «In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente (...) restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi».

Vada avanti, senatore abolisce per i pubblici dipendenti la possibilità di permanenza in servizio oltre il sessantasettesimo anno di età; questa è stata presentata dal ministro Bersani come una misura tendente a favorire un ricambio anche generazionale. Dunque, evidentemente è una norma particolarmente importante che volutamente il Governo un decreto‑legge, cioè un provvedimento che è in sé di straordinaria necessità ed urgenza (altrimenti sarebbe incostituzionale); ha ritenuto che fosse straordinariamente necessario ed urgente

è probabile che sia particolarmente auspicabile un ricambio generazionale anche al suo interno.

questo *stop and go*, questo contraddirsi del Governo, che prima con un provvedimento di straordinaria necessità ed urgenza impedisce ai pubblici dipendenti, dunque anche ai dirigenti del CNR, di rimanere in servizio oltre i 67 anni e dopo pochi mesi cambia idea e con un altro provvedimento di straordinaria necessità

È un fatto davvero notevole. Il senatore Quagliariello ha presentato, con la firma di parecchi altri colleghi, fra i quali quella del sottoscritto, un'interrogazione al riguardo, ma credo sia da sottolineare

che venga prorogato il termine per restare in servizio al 30 giugno 2007 e che sia differita la procedura per attuare i concorsi sempre al 30 giugno, per cui è chiaro che il 1° luglio

poco si fa (mi riferisco naturalmente all'attività del Governo), con conseguente lesione del buon senso, della legge sul conflitto di interessi, di una legge da poco approvata e anche di un minimo di decenza, perché francamente approvare un provvedimento così mirato ad una persona, che è fratello del Presidente del Consiglio, è un'ineleganza che ci si poteva risparmiare.

a questa legge di proroga di termini, che ha la stessa natura delle precedenti e comunque pone sempre il problema della omogeneità

lo stesso provvedimento presenta elementi di pericolosità, di cui voglio fare cenno, sotto il profilo generale adottando il parametro costituzionale. quando si propongono norme con le quali si cerca di intervenire per legge in una controversia fra

(la parte pubblica entra nell'interesse delle parti in causa private) e comunque si cerca di sostituire anche la decisione giudiziale che ormai è in atto. In materia di espropriazione per i fatti del terremoto del 1980 a Napoli, ad esempio, ci troviamo di fronte ad una controversia fra privati cittadini e un consorzio privato di cooperative e lo Stato interviene per dar ragione al consorzio e imporre ai privati limitazioni dei loro interessi generali. Si può fare? È legittimo costituzionalmente? Secondo me no. E poiché,

Questo è un secondo esempio di un modo di legiferare pericoloso che non tiene conto dei parametri costituzionali e dei princìpi contenuti nel nostro Regolamento.

Quali sono gli elementi di pericolosità che determinano una spesa? Non solo, ci sono delle procedure che nella passata legislatura abbiamo posto in essere per garantire sia questi trasferimenti sia una mobilità

che si vedono, in qualche modo, puniti o favoriti, ma senza una motivazione e, soprattutto, senza il rispetto delle regole che la nostra Costituzione

desidero ritornare sull'obbrobrio del comma 5 dell'articolo 1 di questo provvedimento di legge: senatore Malan, poc'anzi, ha evidenziato una delle tante storture di questa disposizione; io ne voglio mettere in evidenza un'altra ancora. La seconda disposizione del suddetto comma introduce un elemento nuovo, cioè la sospensione dell'attività delle commissioni che avrebbero dovuto già da tempo funzionare, in quanto comunque già deliberate prima del 1º gennaio 2007, nonostante quanto prevede la relazione di presentazione del dispositivo in esame

Il bando previsto dal consiglio di amministrazione del CNR è complesso: prevede la costituzione, per ciascuno dei 108 direttori degli istituti, di una commissione, la quale deve esaminare le domande - e proporre al consiglio di amministrazione una terna di candidati idonei a subentrare nella direzione di ogni istituto. Si prevede che il lavoro della commissione richieda almeno tre mesi, perciò se inizierà il 1° luglio, si concluderà il 1° ottobre, al più presto, o anche il 1° novembre. ciascun candidato della rosa verrà sentito dal consiglio di amministrazione - questo è previsto dal bando - e dovrà

il nuovo *set* di direttori dei 108 istituti di ricerca subentrerà - voglio essere ottimista - il 1° gennaio del 2008. Abbiamo, quindi, introdotto un ritardo grave nel funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, assolutamente non giustificato. Il senatore Villone, poc'anzi, nel presentare le proprie controdeduzioni rispetto alla nostra dichiarazione di non costituzionalità del provvedimento in esame e di questa particolare disposizione, ha fatto riferimento al fatto che è in corso un riordino Questa stessa parola - «riordino» - viene citata nella presentazione della relazione di motivazione del provvedimento da parte del Governo.

decreto legislativo n. 127 del 2003, che ha la piena possibilità di gestire con le proprie disposizioni il funzionamento dell'ente. È in di un disegno di legge di riordino, il che, però, non autorizza assolutamente a citare il riordino come se fosse già stato deciso né motiva, perciò, la sospensiva delle procedure concorsuali che ho riferito. In sostanza, tra i tantissimi abusi che questa norma commette, vi è anche l'utilizzo di un presunto dispositivo di legge di riordino che non esiste assolutamente, introducendo così nel funzionamento dell'ente una gravissima disfunzione ed una lesione del principio di responsabilità del consiglio di amministrazione. Ma com'è possibile,

in cui ci si permette di compiere atti abominevoli: certamente questo vuol dire legare le mani ad una gestione che peraltro ha il pieno diritto di essere effettuata a 360 gradi, pretendendo che i gestori i membri del consiglio d'amministrazione continuino ad avere la piena responsabilità. Questo, secondo voi, è un modo corretto di legiferare,

è una bella giornata sia perché è San Valentino, e quindi ci auguriamo che tutti abbiano vissuto un momento positivo con le rispettive metà, sia perché finalmente si vota.

una serie di dubbi dal punto di vista economico. Per esempio, ci piacerebbe sapere dal Ministro dei trasporti dove andranno a finire i circa 67-68 milioni di euro dell'ENAC

a tutti gli italiani dieci euro per le prestazioni specialistiche sul pronto soccorso e se uno ha la sfortuna

che con i soldi dei risparmiatori e degli azionisti vogliono pensare agli affari loro. Vede, Presidente, vi sono alcune Regioni che purtroppo conoscono il pizzo; ebbene, noi conosciamo qualche volta gli emendamenti. Mi riferisco ad un emendamento presentato da alcuni colleghi

che prevede la cessione delle concessioni idroelettriche nel territorio di Trento e Bolzano, fissandone la scadenza al 2010; questo solamente nel territorio di Bolzano,

che solamente l'ENEL, per esempio, ha versato 108 milioni di euro per avere queste concessioni perché il passato Governo ha detto: volete il rinnovo?

Stiamo parlando di un esproprio che non tocca solamente l'ENEL e l'Edison, come aziende in quanto tali, ma anche i risparmiatori. Voi, con un emendamento, andate a toccare la tasca di milioni di risparmiatori.

determinazione e limitazione della norma attualmente vigente, che ha visto anche il favore della Commissione bilancio. Quindi, ci attendiamo un pronunciamento da parte del Governo.

non debba essere invasivo. Se ci sono state delle cartelle pazze, si deve tornare indietro, ma non pensiamo che vi siano cittadini di serie a e di serie b e che quelli di serie b

Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, io interverrò su un punto specifico di questo decreto-legge, in particolare sull'articolo 1, comma 5, il famigerato comma 5. Ebbene, credo che ci troviamo di fronte ad una norma che introduce una sospensione mentre i concorsi sono in svolgimento, secondo una prassi mai prima d'ora attuata in questo Paese. Non era mai accaduto in Italia che un concorso pubblico

credo anzitutto che non sia corretto quanto si è sostenuto e cioè che occorre aspettare l'approvazione del disegno di legge di riforma degli enti di ricerca, che dovrebbe introdurre procedure più trasparenti. Innanzi tutto, perché le commissioni sono composte da commissari di alto livello scientifico, con una reputazione internazionale, spesso sono anche stranieri. Tra l'altro, le modalità di costituzione di tali commissioni per qualche aspetto rispondono persino alle istanze che il ministro Mussi più volte ha sollevato nell'ambito della discussione con le forze politiche anche di opposizione e cioè sono state costituite sulla base di un'indicazione dei consigli scientifici, che hanno proposto dei nomi sulla base, a loro volta, di un elenco di *referee* internazionali:

che non soltanto il decreto, ormai legge, Bersani ha introdotto nel nostro sistema, ma che lo stesso ministro Mussi più volte ha rivendicato per quanto riguarda proprio il governo dei nostri enti di ricerca. Il ministro Mussi più volte ha detto che occorre fare spazio ai giovani, qui invece si procrastina una gerontocrazia. Non voglio fare facile polemica ricordando che uno di questi direttori prorogati è proprio il fratello del Presidente del Consiglio, ma tale provvedimento contrasta anche con le dichiarazioni più volte reiterate di lotta allo *spoils system*. Ebbene, è dall'inizio della legislatura che questo Governo tenta di azzerare i vertici degli enti di ricerca. Aveva cercato di farlo già in occasione del decreto Bersani, poi ci fu quell'emendamento alla legge finanziaria che venne bloccato grazie alla sollevazione di tutto il mondo della ricerca e al duro e forte contrasto dell'opposizione. Evidentemente l'attuale Governo si trova di fronte ad un sistema della ricerca che non riesce ad amministrare e a governare come vorrebbe.

Procederà ad un'ennesima proroga? Continuerà a rinnovare sulla base di proroghe politiche il mandato di quei direttori di istituto, oppure getterà nel caos il CNR? Ecco, di fronte ad un' alternativa di questo tipo ‑ lottizzazione politica o caos ‑ credo che tutte le persone responsabili dovrebbero cassare questa parte del provvedimento, il comma 5 dell'articolo 1, che certamente arreca un grave *vulnus* al nostro sistema e introduce il principio gravissimo, direi eversivo, per cui un Governo con una legge può bloccare un concorso che non riesce a controllare. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che riaffermare quanto ho già avuto occasione di dire nel corso dei lavori della 7ª Commissione: e cioè che questo decreto-legge - cosiddetto mille proroghe - oggi in conversione, adducendo a pretesto la necessità di una serie di proroghe, punta in realtà a bloccare i concorsi nel settore della ricerca. Ciò rappresenta un fatto gravissimo, sul piano politico come su quello più strettamente istituzionale. Anche perché i concorsi rientrano in una procedura amministrativa per cui, se il Governo blocca tale procedura, pone in realtà tutti noi di fronte ad un commissariamento di fatto degli enti interessati. Sotto questo aspetto il mille proroghe getta, fra l'altro, una luce inquietante su un altro provvedimento ancora all'esame della 7ª Commissione: mi riferisco al disegno di legge delega in materia di riordino degli enti di ricerca. Il punto più scandaloso di questo decreto-legge è sicuramente il comma 5 dell'articolo 1, che porta un micidiale attacco all'autonomia e al funzionamento del CNR: ossia del nostro più importante ente di ricerca che, per numero di brevetti, è secondo solo alla FIAT. ricordo qui che, nella relazione al Parlamento sulla gestione del CNR degli anni 2004/2005, la Corte dei conti ha espresso un vivo apprezzamento per i risultati conseguiti dall'attuale consiglio d'amministrazione, sottolineando le conseguenze negative di un eventuale intervento di riordino prima che siano dispiegati gli effetti del decreto legislativo n. 127 del 2003 in fase di applicazione. Parere, questo, condiviso dal consiglio d'amministrazione, dai direttori di dipartimento e dalla comunità scientifica interna ed esterna all'ente, la quale ha inviato al riguardo una lettera firmata da 700 ricercatori al Ministro dell'università e della ricerca. Ricordo altresì che, sempre nella suddetta relazione, la Corte dei conti osservava come gli attuali direttori di istituto - che saranno tra i beneficiari del mille proroghe, se questi verrà approvato sono proprio coloro che hanno opposto resistenza al cambiamento e all'azione di rinnovamento generazionale dei direttori di istituto del CNR. E, del resto, tale ostilità al cambiamento, da parte dei direttori di istituto più anziani (per età e carica), è confermata dalla presentazione di ricorsi al TAR del Lazio per l'annullamento dei bandi, che sono ancora in attesa di decisione sul merito dopo l'infruttuosa richiesta di sospensiva dei ricorrenti. Ma tornando al famigerato comma 5 dell'articolo 1, non posso non rilevare la falsità della motivazione enunciata nella relazione governativa al decreto-legge, la quale recita: «La norma è necessaria al fine di consentire la prosecuzione della funzionalità del Consiglio nazionale (...). Allo stesso tempo, l'eventuale rinnovo degli incarichi di direzione potrebbe risultare incoerente con l'assetto dell'ente all'esito della fase di riordino». ripeto, tutto ciò è falso. Perché il 20 dicembre 2006 gli incarichi erano già stati prorogati fino al 30 giugno 2007 dal consiglio di amministrazione, impegnato dal 2004 ad applicare con successo il decreto legislativo n. 127 del 2003 di riordino del CNR. Perché le procedure concorsuali per la selezione dei direttori di istituto non sono solo già definite, ma sono anche in fase di espletamento a seguito dei bandi internazionali con termini già scaduti? Perché non esiste

rinvia semplicemente *sine die* lo *status quo*, affermando, in definitiva, che si vuole sospendere l'applicazione della legge vigente, per meglio applicare in futuro una potenziale norma di legge, peraltro totalmente *in fieri*. Questo è quanto meno un bizzarro modo di procedere. La verità, invece, è che è proprio il comma 5 dell'articolo 1 a pregiudicare la funzionalità del CNR, tanto sul piano dell'autonomia che sul piano dei contenuti. Sul piano del rispetto dell'autonomia, poiché l'intervento proposto ha un impatto negativo sul sistema della separazione delle responsabilità. Approvando il decreto, infatti, il consiglio d'amministrazione del CNR verrà deresponsabilizzato e le sue funzioni saranno invase dal Governo, con il risultato che esso non potrà più essere chiamato a rispondere dei risultati. Sul piano dei contenuti, infine, perché blocca, nonostante i risultati conseguiti, il cambiamento in atto al CNR. Ricordo, in proposito, che il consiglio d'amministrazione, insediato nel 2004, ha approvato il nuovo quadro organizzativo e regolamentare; ha ridotto il numero, integrandole tra loro, di quelle strutture scientifiche con autonomia di spesa che erano frammentate; ha costituito tutti gli organi di consulenza scientifica e di valutazione; ha istituito 11 nuove strutture dipartimentali con compiti di coordinamento, come previsto dalla normativa vigente, selezionandone i direttori; ha, infine, avviato l'ulteriore riorganizzazione della rete degli istituti distribuita sul territorio e ancora con forti duplicazioni. Sempre sul piano dei contenuti, perché impedisce il ricambio nella direzione degli istituti. La maggior parte dei direttori scaduti dirige le strutture da un numero considerevole e ininterrotto di anni (alcuni addirittura da più di 30 anni!), pur in presenza di un limite di due mandati, aggirato però negli ultimi anni con riorganizzazioni prevalentemente di facciata, limitate al semplice cambio di denominazione delle strutture stesse. luogo, sempre sul piano dei contenuti, perché il blocco del ricambio è in controtendenza rispetto alle scelte generali sulla pubblica amministrazione. La norma del decreto-legge è, di fatto, una norma di deroga immotivata a quei limiti di età, relativi al conferimento di incarichi che comportano funzioni dirigenziali, posti proprio dal cosiddetto decreto Bersani-Visco per tutta l'amministrazione pubblica (ivi inclusi gli enti di ricerca). Con tale norma, ad esempio, circa 30 dirigenti del CNR, che al 31 dicembre 2006 hanno compiuto 67 anni, continueranno a rivestire l'incarico di direttore di istituto. Rimarrà in carica anche il più anziano di questi, il quale ha compiuto 79 anni! Quarto, sempre sul piano dei contenuti, perché impedisce un aumento di funzionalità derivante dall'effettivo esercizio del tempo pieno. La nuova norma consentirà infatti a professori universitari a tempo pieno di mantenere ulteriormente l'incarico simultaneo di direzione di un istituto del CNR, nonostante questa simultaneità sia in contrasto con la normativa vigente. 30 su 80 dei direttori di istituti prorogati continueranno perciò ad avvalersi di un meccanismo di deroga alle norme che obbligano i professori universitari a mettersi in aspettativa; meccanismo, questo, che faceva parte del precedente quadro regolamentare e che fu eliminato dal decreto legislativo n. 127 del 2003, con la possibilità di essere mantenuto solo transitoriamente. Infine, sempre sul piano dei contenuti, perché causerà certamente una situazione di grave difficoltà gestionale il 1° luglio, quando scadrà la proroga stabilita dal decreto-legge, senza che sia stato possibile individuare i nuovi direttori di istituto. In concreto, la proroga prevista da questo decreto-legge determina - rispetto alla proroga per delibera del consiglio d'amministrazione del CNR - un azzeramento dei vincoli sui limiti di età e un rinvio dell'entrata in vigore della obbligatorietà del tempo pieno. Sono due effetti nettamente in controtendenza rispetto a questioni molto attuali, particolarmente sentite dall'opinione pubblica, la quale chiede ringiovanimento dei vertici pubblici e opportunità per i giovani con riferimento specifico al mondo dell'università e della ricerca, così come chiede, altresì, di eliminare i doppi incarichi. La norma inserita nel decreto-legge in corso di conversione presenta inoltre diversi profili di incostituzionalità, oltre a sostanziare un'evidente interferenza del potere legislativo nelle scelte e negli atti amministrativi di un ente pubblico autonomo (interferenza, questa, ancor più censurabile in quanto si tratta di ente a carattere non strumentale con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, protetta dall'articolo 33 della Costituzione), tanto più che sono del tutto assenti i presupposti di straordinarietà, necessità ed urgenza dell'intervento per decreto-legge, richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Non sono sostenibili né la necessità, né l'urgenza visto che, come già accennato, il consiglio d'amministrazione del CNR aveva disposto una proroga precedente all'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto-legge in questione. La norma configura pertanto una specie di legge provvedimento, ammessa nel nostro ordinamento solo in via eccezionale e sempre in presenza di situazioni particolari di interesse generale. Nel caso di specie, purtroppo, non si ravvisa alcun interesse generale, bensì solo un consolidamento di singole situazioni personali. di singole situazioni personali. Vedete, onorevoli colleghi, la definizione di mille proroghe, affibbiata al decreto-legge in corso di conversione dal dibattito politico, rimanda per analogia ed assonanza alla figura del millepiedi. Ma, data la logica che ispira tale provvedimento, sarebbe forse meglio parlare di un mille mani: mille mani libere del Governo a danno dell'autonomia della ricerca, per la realizzazione, peraltro, di un disegno di mera conservazione, teso a garantire i supergarantiti di sempre e a rendere ancora più inamovibili gli eterni inamovibili. un disegno di chiusura corporativa a vantaggio di una certo potere accademico. Un contentino ad alcune baronie universitarie e a qualche clientela elettorale. A danno dei giovani e del bisogno di cambiamento e innovazione del mondo della ricerca. A danno, insomma, dell'Italia e del suo futuro.

esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti del Governo, esprime, per quanto di propria competenza e ad eccezione degli articoli 2 e 6, parere non ostativo, ai seguenti presupposti: che l'articolo 1, comma 1, non abbia implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato né dei bilanci degli Atenei, risultando volto alla salvaguardia della programmazione dei fabbisogni universitari; che, con riferimento all'articolo 2, comma 3, non si registrino effetti finanziari negativi in termini di minori entrate sul bilancio dell'anno 2006; - con riferimento all'articolo 2, comma 4, che vi sia l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste a copertura della disposizione; che siano esclusi effetti finanziari negativi associati all'articolo 3, comma 3; - con riferimento all'articolo 3-*bis*, risulti limitata la platea dei beneficiari delle agevolazioni previste e risulti sufficientemente congruo il relativo limite di spesa; in relazione all'articolo 4, comma 1, sia fatta salva la realizzazione degli obiettivi di risparmio pubblico previsti dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; che l'articolo 6, comma 2, disponga una mera proroga temporale e non rechi alcuna ulteriore autorizzazione di spesa relativamente agli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; - che l'articolo 6, 4, non comporti oneri aggiuntivi, operando la disposizione nell'ambito delle somme già stanziate per i programmi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286. Esprime, poi, parere contrario sull'articolo 6, comma 5, nonché parere non ostativo sugli articoli 2 e 6, alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che al comma 3 dell'articolo 2, le parole: «pari a» vengano sostituite dalle altre: «valutato in»; - che dopo il comma 3 dell'articolo 2 venga aggiunto il seguente: «3-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. che venga soppresso il comma 8 dell'articolo 6; - che al comma 8-*quater* dell'articolo 6 la parola: «determinato» venga sostituita dall'altra: «valutato»; che al comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 le parole: «pari a» vengano sostituite dalle altre: «valutato in»; - che dopo il comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 venga aggiunto il seguente: «8-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-*ter* e 8-*quinquies*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.16, 1.38, 1.39, 1.9, 1.37, 1.40, 1.46, 1.41,

6.49, 6.50, 6.8, 6.73 (limitatamente al capo verso 8-*sexies*), nonché parere contrario sugli emendamenti 6.9, 6.73 (limitatamente al capoverso capoverso 8-*septies*). Esprime altresì parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, anche sugli emendamenti 2.501, 2.500, 3.500, 3.501, 4.0.500, 6.501, 1.800, 6.0.380 (limitatamente al comma 4), 1.150 e 1.901. Esprime altresì parere contrario in ordine all'emendamento 6.0.380 (limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 5) e sull'emendamento 1.900. Esprime, infine, parere non ostativo sull'emendamento 1.31 nel presupposto che non abbia implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato né dei bilanci degli atenei, nonché sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte di seguito indicate per le quali il parere è reso a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'emendamento 6.55 vengano inserite le seguenti parole: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili» - che all'emendamento 6-bis.0.100 le parole: "all'adozione" vengano sostituite dalle altre: "all'entrata in vigore"». bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sugli emendamenti 6.800, 1.150 (testo 2) e 6.73 (testo 2) limitatamente al comma 8-*septies*. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.380 (testo 2) a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano soppresse le parole: "sino al completamento dei relativi interventi". Esprime, poi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.73 (testo 2) limitatamente al comma 8-*sexies*. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2) a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le parole: "in materia di mobilità" siano sostituite dalle seguenti: "in materia di trattamento economico del personale in mobilità".

il Governo avrebbe presentato finalmente le relazioni tecniche, che da due giorni sto richiedendo per fare in modo che si possa formulare un parere documentato. Mi dispiace, quindi, ma le chiedo dieci minuti di sospensione per poter riunire la Commissione. In caso contrario, sarei costretto

tenuto conto della complessità dei pareri di cui ho dovuto dare lettura e della difficoltà che, credo, abbia trovato sul suo percorso la Commissione, temo di non poter accedere alla sua richiesta. Mi segnalerete, nel corso dell'esame, gli emendamenti del resto, credo che di queste riformulazioni ce ne saranno diverse, così a fine seduta le affrontate tutte in un'unica soluzione e procediamo finalmente con i nostri lavori.

più volte modificato e l'ultima volta modificato con il decreto cosiddetto Bersani del luglio scorso. Si tratta di questo: i medici che esercitano negli ospedali pubblici possono, in alternativa allo svolgimento di un'attività a tutti gli effetti esterna rispetto all'ospedale, svolgere un'attività di carattere libero professionale, ma all'interno dell'ospedale stesso; all'interno da un punto di vista, in teoria, anche fisico, cioè intramurario, cosiddetto *intramoenia*. Tuttavia, poiché gli ospedali hanno già difficoltà notevoli a garantire un'assistenza adeguata e strutture adeguate e in molti casi non riescono neppure a garantire strutture adeguate per l'attività a tutti gli effetti pubblica, da diversi anni sono proroghe e si è data la facoltà a quei medici di esercitare anche al di fuori delle strutture ospedaliere, ma diremo così - per conto dello stesso ospedale dal quale dipendono. All'ospedale va una percentuale anche rilevante di quanto i medici incassano.

Francamente, non vedo ragione per impedire il proseguimento di questo tipo di attività. Tuttavia, il decreto cosiddetto Bersani ha stabilito che entro, e non oltre, il 31 luglio 2007 tutte le strutture ospedaliere dovranno adeguarsi in modo da consentire ai medici di esercitare questa attività, che, lo ricordo ancora,

In Commissione sanità sono state fatte numerose audizioni. Tutte le persone audite hanno concordato nel dire che è impossibile che entro il 31 luglio di quest'anno si completino questi adeguamenti.

Riterrei più giusto che le strutture sanitarie pubbliche investissero le risorse finanziarie di cui dispongono, che per loro natura sono limitate, nel migliorare le strutture che

termine che non sia completamente impossibile rispettare. Io ho proposto quello del 31 dicembre 2010, lasciando ad altra sede la discussione sull'opportunità in assoluto di arrivare a questa limitazione.

si lede il diritto di autonomia dell'ente di ricerca; ai sensi dell'articolo 97, perché si lede il dovere di imparzialità e di buona amministrazione della pubblica amministrazione che ha il legislatore quando legifera;

lesivo dell'attività dell'ente e delegittimante l'attività del consiglio d'amministrazione. Chiedo veramente che i *senatores,* che sono tutti *boni* *viri,* non diventino *Senatus* in questa particolare votazione.

si propone di consentire al CONI di portare avanti tutte le procedure relative al trasferimento di personale in seguito alla privatizzazione dell'ente,

in particolare i processi di mobilità relativi alle federazioni. Speriamo di aver trovato una formula accettata dal Governo e dal relatore e chiediamo l'approvazione di questi emendamenti che riguardano un ente a tutti noi caro, che si occupa dell'organizzazione dello sport.

la mobilità del personale di CONI Servizi Spa verso la pubblica amministrazione. Naturalmente, sono favorevole alla soluzione individuata e attendo il parere del rappresentante del Governo e del relatore per esprimere la successiva dichiarazione di voto.

Il primo criterio generale è quello di esprimere un parere contrario su tutti gli emendamenti che tendono a sopprimere, in tutto o in parte, la norma così come trasmessa dalla Camera. Il secondo criterio è quello di tener conto, ovviamente, delle opinioni espresse dalla Commissione bilancio, sia quelle *ex* articolo 81, sia quelle che non si riferiscono all'articolo 81 della Costituzione. Questo, naturalmente, per quanto riguarda il maggior numero possibile di materie. peraltro, alcuni punti su cui esprimerò un parere favorevole, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere difforme, ma, ripeto, non *ex* articolo 81 della Costituzione. poi di esprimere pareri favorevoli su emendamenti fondati, assentiti, sui quali c'è una pluralità di proposte che provengono da senatori appartenenti a diversi Gruppi parlamentari in modo da tenere conto anche di questo criterio molto importante. Detto questo, passo all'espressione dei pareri all'articolo 1.

parere è favorevole all'emendamento 1.1 (testo 2), ma riformulato secondo le raccomandazioni della Commissione bilancio, la quale ha

per la disamina di ulteriori emendamenti, presentati, naturalmente, sotto la

con l'occasione di riformularli - e che si tratti di vere e proprie ripresentazioni è dato dalla circostanza che la Commissione bilancio debba riunirsi per riprenderli in esame - mi pare che non sia

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sugli emendamenti 6.800 e 1.150 (testo 2) e 6.73 (testo 2) limitatamente al comma 8-*septies*».

si troveranno ad avere 56.000 medici che non possono lavorare (medici che sia che lavorino privatamente, sia che operino

a far sì che le assunzioni siano prioritariamente finalizzate al completamento degli organici delle sedi sottodotate e, per il futuro, a valutare l'opportunità di effettuare graduatorie regionalizzate. Purtroppo oggi si registrano assunzioni in determinate Regioni e, dopo poco tempo,

invito il Senato a considerare l'emendamento 1.900 con attenzione. I giudici onorari aggregati hanno dato prova di grande capacità ed hanno contribuito sensibilmente alla definizione di molti processi stralcio. Il carico oneroso della giustizia civile è stato ridotto, anche se in maniera sensibile, grazie al loro impegno. Far cessare la loro attività mi pare confligga con le esigenze di una celere trattazione dei processi, soluzione auspicata anche qualche tempo fa in maniera molto enfatica, devo dire, dal Ministro della giustizia. Allora, invito il Senato a considerare la possibilità di prorogare le funzioni dei giudici onorari aggregati proprio per consentire che il loro impegno vada avanti ulteriormente con sensibili vantaggi per la giustizia. Presidente, chiedo al senatore Valentino di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 1.900. Come anche il Ministro della giustizia qui presente ben sa, non costa nulla; in ogni caso verrebbero nominati altri, ma si disperderebbe un patrimonio di esperienza che invece è utilissimo e consente di far funzionare un po' meglio (o meno peggio) la macchina della giustizia, che, peraltro, mi consenta il Ministro, è stata ulteriormente falcidiata dalle azioni di questo Governo, non ultimi il decreto Bersani e la legge finanziaria. Quindi, sarebbe veramente utile che questo emendamento fosse approvato dall'Assemblea e

l'emendamento 3.2. L'articolo 3 comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, prevede disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastutturali e lavori in edilizia. In pratica, esso riconosce efficacia agli accordi in ordine alle indennità da corrispondere ai soggetti coinvolti nei procedimenti di espropriazione di cui alla legge n. 219 del 1981 per il terremoto, anche quando il decreto di espropriazione per pubblica utilità non sia stato emanato nei termini. In materia esistono nutrite critiche che ritengono tale comma estraneo al campo operativo del mille proroghe laddove, ancorché riguardi un atto di natura pubblica, non prevede alcuna proroga in termini. Addirittura c'è chi ritiene che l'emendamento in oggetto contrasti con il consolidato orientamento giurisprudenziale. Molti giudici infatti riconoscono legittimo il diritto degli espropriati, seppur firmatari di «concordamento dell'indennità», di conseguire anche il risarcimento del danno per giunta commisurato al valore di mercato del cespite. Invero, al di là delle critiche e delle opinioni discordanti, il dato di fatto è che la norma, per quanto perfettibile, esiste e che il mille proroghe ci offre la possibilità di intervenire. In tal senso, la *ratio* del presente emendamento che si pone quale atto mediativo per salvaguardare le parti interessate. In particolare, l'intervento in oggetto è a vantaggio di tutti i cittadini coinvolti nei contenziosi che, seppur non potranno percepire dalle imprese concessionarie quanto ritengano di spettanza, almeno saranno esonerati dal pagare le spese giudiziarie poste viceversa a carico dello Stato.

anzitutto andrebbe fatta una precisazione per quanto riguarda la materia trattata dall'articolo 3, che si riferisce a degli espropri, avvenuti nel 1981, di piccoli appezzamenti agricoli ai fini della ricostruzione dopo il terremoto del novembre del 1980.

sostenendo che vada ritenuta inefficace la subentrata norma di proroga quando, per effetto della scadenza del termine originario, si sia già verificata la cosiddetta accessione invertita. Questo sostanzialmente significa che, non essendo più legittima la proroga, dalla scadenza della proroga al momento attuale l'occupazione viene ritenuta illegittima. Questo viene riconosciuto, tanto che nella relazione si legge che tutto il periodo di occupazione, scaduto il termine originario, va qualificato come occupazione illegittima e, di conseguenza, viene ritenuto necessario il pagamento di risarcimento del danno e l'indennità, a seguito dell'accessione invertita, e perdono quindi efficacia gli atti di concordamento bonario dell'indennità. Questo significa, in sostanza, che tutti quanti i proprietari legittimi di questi appezzamenti di terreno hanno fatto ricorso in tribunale per chiedere il risarcimento del danno per occupazione illegittima e significa altresì che il Governo con questo articolo vorrebbe fare, non già una proroga, ma una sanatoria di proroghe illegittime, che sono state ritenute illegittime della Suprema corte, il che credo sia quanto meno incostituzionale. Si interviene così su 180 cause già in atto, che stanno andando in giudizio e, di conseguenza, ai singoli cittadini che hanno fatto ricorso di avere un giusto processo e di ottenere quello che la legge sostanzialmente sancisce. C'è però un elemento più grave: in realtà l'articolo 3 viene giustificato

del CIPE del 1990 e un parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli che dicono chiaramente che il responsabile di questa illecita occupazione non è lo Stato, bensì il consorzio delle cooperative di costruzione che era titolare dell'esproprio. Le 180 cause a cui si fa riferimento non sono contro lo Stato o la pubblica amministrazione, ma contro un soggetto privato che è un consorzio delle cooperative. Di conseguenza, l'articolo 3 non va ad impedire un danno per l'erario dello Stato, ma interviene anzitutto su una causa tra due soggetti privati (privilegiandone uno, ossia un grosso consorzio che ha grandi appalti e grandi legami con le pubbliche amministrazioni, contro dei singoli cittadini), e va poi praticamente a giustificare questo atto di interferenza con l'operato della magistratura addossando allo Stato la responsabilità di questa occupazione abusiva. Io ritengo - il relatore oggi in 1ª Commissione sembrava pensarla alla stessa maniera - che, se non si

che ci sono già 180 procedimenti in atto che stanno andando a conclusione e, grazie alle sentenze della Suprema Corte e al parere dell'Avvocatura dello Stato, andranno a favore dei singoli cittadini. Non credo che il Parlamento possa approvare una legge

imprenditori agricoli, di 180 piccoli proprietari a cui, in questo caso, verrebbe negato anche il diritto costituzionale di un equo processo.

che, con l'introduzione dell'*ex* articolo 12, trasformato in finanziaria, una sentenza del tribunale di Genova ha invitato il Governo a sospendere qualsiasi iniziativa nel merito; non solo, ma ha chiesto alla Corte di giustizia europea

sull'ordine del giorno che verrà presentato da alcuni colleghi in sostituzione della parte non assentita dalla Commissione dell'emendamento originariamente presentato.

sulla necessità che venga accolto questo emendamento, che non rimette in discussione l'entrata a gamba tesa che il ministro Di Pietro ha inteso fare con la norma della finanziaria con cui ha azzerato le concessioni in essere. Con un provvedimento di legge, si è cancellato un atto che le parti contraenti hanno liberamente sottoscritto. Decideranno i tribunali se è legittimo, oppure no. Con tale emendamento si intende solo differire nel tempo la decorrenza di questa norma assurda.

pacatamente che tipo di ricaduta avranno queste norme. Faccio presente che, dal momento in cui il Parlamento ha approvato questa norma, nel settore regna la paralisi, gli investimenti sono

non si applicano nei casi di pendenza di procedimenti giudiziari relativi ai beni oggetto dell'esproprio e alla procedura di esproprio».

per la struttura di coordinamento che si è fatta sulle scuole senza toccare l'impianto che si è determinato con l'emendamento in finanziaria. Quindi, vorrei chiarire ai colleghi che se ne preoccupano che non si tocca la struttura della norma, ma si determinano solo le condizioni che cercano di evitare l'incertezza nelle scelte individuali di passaggio, perché ci sono passaggi di personale. Vorrei rassicurare sul fatto che si tratta di modifiche dalla portata assolutamente limitata che non incidono sull'impianto.

con questo emendamento si sta creando una grave disparità territoriale. È assurdo che nelle Province di Trento e Bolzano i concessionari di energia idroelettrica non godano più della proroga che garantirebbe i loro contratti. Chiedo, qualora questa maggioranza decidesse di votare a favore dell'emendamento in questione, che il relatore e il Governo prendano in considerazione l'eventualità di risarcire

centinaia, migliaia di risparmiatori e di azionisti di aziende quotate in borsa (e mi riferisco all'ENEL e ad Edison).

La norma del decreto Bersani aveva ridotto la proroga delle concessioni fino al 2030, per quanto riguarda l'ENEL.

lo Stato, allora, lo ha eliminato, a fronte di un'adeguata proroga delle concessioni in essere (ricordo che negli altri Stati membri la durata media del regime di concessione è fino al 2050).

serie di provvedimenti, in primo luogo economici, per cui la proroga è subordinata ad interventi di ammodernamento e sugli impianti sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza:

in questo provvedimento, qual è l'utile per le casse dello Stato? Zero! Sarebbe stato possibile, eventualmente, formulare un emendamento con il quale chiedere la revoca a fronte di ciò o fissare una proroga onerosa.

quindi ad influire sul bilancio di aziende quotate in borsa per centinaia di milioni di euro. In questo modo non facciamo un dispetto al signor Conti o al signor Quadrino,

Il problema allora nacque distinguendo l'interesse nazionale da quelli prettamente locali e operando una distinzione tra le grandi e le piccole derivazioni. Già dall'epoca le piccole derivazioni vennero lasciate alle Province autonome; rimase in capo allo Stato, *ergo* alla concessionaria di Stato, l'ENEL, la gestione delle grandi derivazioni e della produzione che fino a poco tempo fa giaceva sotto monopolio nazionale tramite l'Ente nazionale energia elettrica.

la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica; una volta approvato a livello nazionale il Piano energetico locale, *ergo* provinciale con tecnici - indubbiamente dell'ENEL - e con tecnici del Ministero; una volta attivato un Comitato misto ENEL-Provincia in quanto il sistema di produzione e distribuzione non può essere parcellizzato ma deve funzionare come sistema armonico, scatteranno agli enti locali, *ergo* a queste società delle Province, le attribuzioni previste nel decreto. Si parlava distintamente di produzione, trasporto e distribuzione in quanto molto più facile era entrare entrare nei due secondi settori; per quanto concerne la produzione, vi è stato un ritardo, di fatto, perché esistevano i predecessori, i concessionari che vantavano indubbiamente il diritto a mantenere la concessione fino alla scadenza, avendo del resto pagato allo Stato gli oneri per poterla mantenere. Pertanto si sancisce questo subentro a livello locale. Il primo decreto Bersani del 1999 scardina un tantino il tutto perché stabilisce, *ergo* decreta, la proroga delle concessioni in essere. Va anche contro un precedente impegno nei confronti delle autonomie locali, che giustamente interpellano la Corte costituzionale perché rivendicano le proprie competenze e i propri diritti, cioè il rispetto dello Statuto e dei decreti attuativi delle norme statutarie. Di più: il decreto Bersani viene punito da una procedura di infrazione perché la stessa Commissione europea non consente più le proroghe automatiche in quanto

condivido? Soltanto che ENEL o i concessionari che hanno una lunga o rinnovata concessione la portino fino al termine (2030, 2035, 2040);

che una materia agognata ed importante, economicamente strategica, potesse passare dallo Stato alle Regioni. Vorrei che tutte le Regioni potessero chiedere ed ottenere che la materia energetica fosse non più sotto le mani delle concessioni statali, ma sotto egida delle singole comunità locali o delle Regioni.

del 1946 tra l'Austria e l'Italia), le travagliate storie dopo il 1946 fino al 1972, le lotte per un nuovo Statuto di autonomia e, dal 1972, in poi le lotte per l'attuazione dello stesso Statuto di rango costituzionale. Naturalmente, con quest'ultimo si è creata una situazione di forte distensione che garantisce una pacifica convivenza in questo territorio la cui specialità è proprio frutto della storia dei patti internazionali, non può essere È inutile che poi, ogniqualvolta si parla di tali diversità, si afferma che tutto il territorio dev'essere uguale; siamo molto d'accordo su questo aspetto, non però nel senso inverso di ridurre quanto con grande fatica siamo riusciti a raggiungere.

Siamo d'accordo, possiamo anche fare da battistrada per portare tutti a un livello più vicino alla gente, perché l'autonomia, in fin dei conti, non è altro che gestire la politica più vicino alla gente. Fatta questa premessa politica, e ringrazio soprattutto per questo sostegno venuto dal collega Divina, che ha compreso e vissuto tutto ciò, vorrei solo ricordare la situazione giuridica

alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale

*(Aut)*. Poi, in esecuzione di ciò, la legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, ha previsto ha previsto una procedura speciale. Ma cosa è accaduto su base nazionale? Il decreto Bersani del 1999

In base a questo la Provincia ha disciplinato la materia con legge provinciale e ha bandito la gara

si adegua alla materia, però «salvi gli effetti di cui alle procedure di rilascio, proroga e rinnovo delle concessioni (...)». E questa legge provinciale è in vigore perché il Governo non l'ha mai impugnata. Pertanto, dal punto di vista giuridico

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi chiedo un attimo di attenzione, perché stiamo entrando su un terreno molto delicato su cui possiamo scivolare e farci male. Ho la vaga impressione che a volte non abbiamo una piena consapevolezza della gerarchia delle fonti di diritto all'interno dell'Unione Europea, perché se l'avessimo, signor Presidente, forse gli uffici del Senato non avrebbero ricevuto questo emendamento; forse il Governo avrebbe dovuto fare un esame di compatibilità europea per esso e avrebbero dovuto concludere che, essendo incompatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Esecutivo, esso è irricevibile, o quanto meno il Governo avrebbe dovuto esprimere un parere negativo. Non so chi mi sta ascoltando dai banchi del Governo, ma sarebbe interessante se qualcuno lo facesse, perché stiamo per infilarci, temo, dentro una procedura di infrazione europea da cui potremmo uscire molto malconci. E per una maggioranza che a suo tempo, quando era minoranza, non perdeva occasione per sottolineare la sua vocazione europeista e per attaccare la maggioranza di allora, oggi diventata minoranza, dicendole che non era abbastanza europeista, sarebbe il terzo, il quarto o il quinto *autogol*, dopo una serie di altre vicende che ci stanno facendo fare, a livello europeo, una pessima figura. Lo dico perché la materia delle concessioni è stata oggetto di un inizio di procedura di infrazione: di una domanda di informazioni prima poi di una lettera di messa in mora. Abbiamo trattato e raggiunto delle soluzioni concordate con la Commissione europea, con il commissario Bolkestein, allora titolare del settore. Ma possiamo oggi intervenire su cose che erano già state risolte, alterando un accordo raggiunto e creando le condizioni perché si riapra, questa volta senza possibilità di bloccarla,

di votare senza avere piena coscienza di quello che sta votando. Ho il forte dubbio che votare a favore di questo emendamento significhi mettere l'Italia nelle condizioni di aprire un contenzioso da cui usciremo male

non solo ci avviamo a prendere un «bagno» terribile in sede europea, ma per di più rischiamo di far rimettere in discussione l'accordo che abbiamo raggiunto su tutte le altre concessioni.

Presidente, intervengo in dissenso per evidenziare come abbiamo fatto male, o hanno fatto male, a non modificare il titolo V della parte II della Costituzione quando si è trattato di competenze in materia di energia. È incredibile che il sistema dell'energia possa essere gestito in modo territoriale, creando un grosso problema al territorio nazionale. A un certo punto la Regione siciliana domani mattina, sulla stessa logica del collega che ha parlato, potrebbe togliere le concessioni alle centrali ENEL di Termini Imerese, di Priolo e di Milazzo, tenendo all'oscuro tutto il Meridione

la condizione che viene introdotta per le Province di Trento e Bolzano, per costante giurisprudenza costituzionale, non può che essere introdotta anche per le altre Regioni a Statuto speciale che ne facciano richiesta. Si verrebbe ad introdurre un grave scompenso dal punto di vista economico, in quanto i ritorni economici, che in questo momento fanno capo a certi concessionari, nel momento in cui una gara viene introdotta

potuta fare perché non era stata osservata la successione delle norme, e quindi la gerarchia delle fonti, alle quali il senatore Peterlini si riferisce. Il Governo dovrebbe ben stare attento perché ciò di cui stiamo parlando ha una rilevanza economica di alcuni miliardi di euro. Dalle stesse dissertazioni fatte dal senatore Peterlini, soltanto per Trento e Bolzano significherebbe una trattazione economica di circa un miliardo di euro, ma, anche per quello che ha detto il senatore Antonio verrebbe ad essere molto più amplificata, ad esempio, nella Regione siciliana che, come sappiamo, produce il 30 per cento dell'energia elettrica che si produce in Italia. Il parere favorevole dato dal Governo mi sembra quanto meno di una leggerezza sconfortante e di una disinvoltura che mi lascia

È una riforma che ha bisogno di una procedura comunitaria; se fissiamo la scadenza al 30 marzo, difficilmente la si potrà concludere.

sappiamo essere necessarie per rendere competitivo l'autotrasporto del nostro Paese.

l'emendamento 6.52, confortato anche dal parere della Commissione igiene e sanità, che aveva immesso in appunto anche la questione nel deliberato il relazione a questa legge. Il governo Berlusconi, con il decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 19, ha recepito nella legislazione nazionale la direttiva europea 2001/83/CE. Tale recepimento risulta particolarmente restrittivo per quanto concerne i farmaci omeopatici ed antroposofici, la cui vendita in Italia corre il rischio di essere penalizzata a causa dei criteri restrittivi, introdotti nel succitato decreto, assolutamente arretrati rispetto alle norme vigenti in altri Stati dell'Unione. Per i farmaci omeopatici e antroposofici, infatti, l'articolo 3 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 185, ha disposto: «L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale omeopatico è rilasciata con procedura semplificata di registrazione», mediante decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 6. Tale autorizzazione, disposta dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto, più volte reiterata, è stata prorogata al 31 dicembre 2008 con la legge del 27 dicembre 2002, n. 289 I medicinali omeopatici ed antroposofici, regolamentati alla data del 6 giugno 1995 ed attualmente in commercio, sono valutati in un numero di circa 50.000 specialità. Ciò conferma la loro validità, nonché l'interesse dei nostri concittadini nei confronti di queste forme di medicina. Va, inoltre, fatto rilevare che la richiesta di una idonea documentazione tecnico-scientifica, necessaria per l'autorizzazione alla vendita, ne dimostra ulteriormente la scientificità. Purtroppo, Purtroppo, nel nostro Paese, malgrado la legislazione ed i fatti su esposti, non è stata costruita una attenzione sufficiente nei confronti delle medicine non convenzionali, al punto che non esiste ancora una documentazione amministrativa adeguata per la presentazione di queste domande. II Governo francese, che pure nel 2000 aveva già fornito un modello di documentazione per presentare le domande di autorizzazione, a seguito del recepimento della direttiva comunitaria, ha fissato il termine ultimo per la proroga

Concludo dicendo che mantengo l'emendamento 6.52, sia per la valenza in sé, sia perché è nell'interesse della nostra economia, sia perché vi è una grave disattenzione verso questo settore che interessa moltissimi cittadini, tant'è vero che anche nell'ultimo

Negli anni si è registrata una gestione aziendale condizionata dai *diktat* di Forza Italia, ma sperperare 20.000 euro per una pubblicazione di due intere pagine a colori è una vergogna, un'offesa alle tasche dei contribuenti, alle istituzioni rappresentate dalla GESAP, come il Comune di Palermo, il Comune di Cinisi, la Provincia di Palermo e la camera di commercio, e all'esigua minoranza di privati. Nella mia interrogazione ribadisco la necessità di controllare, non solo l'operato, ma anche l'utilizzo delle risorse. La GESAP non può essere la succursale di Forza Italia, realtà acclarata dalla presenza ai ruoli apicali di dirigenti dello stesso partito. Ecco perché, fermo restando le valutazioni che il Ministro farà sulla convenzione, ritengo necessario che si proceda ad una attenta analisi sugli sperperi e sui disservizi che spesso sono stati evidenziati e che gravano sui passeggeri e sui lavoratori della struttura, il cui impegno è encomiabile, disservizi che si manifestano da anni e non solo in quest'ultimo periodo. Basta quindi agli sprechi e alle aziende lottizzate. Nulla contro i presentatori di un atto ispettivo che rientra nelle prerogative dei colleghi, i quali, sono certo, converranno con me che la spesa sostenuta non rientra nei princìpi di una oculata gestione di una azienda a prevalente capitale pubblico.

stata inviata il 1° maggio del 2005, ossia un anno e undici mesi fa, di cui solo otto sotto il Governo Prodi. Perché non si lamentava prima? Perché la GESAP non ha assunto una iniziativa così clamorosa e costosa

La seduta è ripresa. Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Roberto Castelli

La vittima della calunnia è una persona che afferma essere membro dei servizi segreti russi e il reato di calunnia è stato constatato oltre un anno dopo che la cosiddetta calunnia sarebbe avvenuta. Ho presentato

un anno prima, è veramente un fatto che, se non implicasse la libertà di un uomo, sarebbe soltanto grottesco; così, invece, arriviamo al vergognoso.

informazioni non sono mai state verificate dalla magistratura, che non ha mai tentato di ascoltare Alexander Litvinienko nei 12 mesi successivi alle informazioni rese da Scaramella al commissariato di Napoli

che quanto prescrive la Costituzione, cioè che le intercettazioni telefoniche o di altro tipo di corrispondenza possono essere disposte ai parlamentari soltanto con l'autorizzazione della rispettiva Camera, può essere tranquillamente eluso, sottoponendo ad intercettazione

il presidente Marini ha riferito le sue preoccupazioni. sue preoccupazioni. Penso che il ministro Mastella, che è stato qui disciplinatamente tutto il pomeriggio per votare la proroga dei termini per consentire a Franco Prodi di restare a capo di un dipartimento del CNR,

estremamente discutibile che un Ministero metta sotto controllo il Parlamento. Eventualmente sarà il Parlamento a controllare l'Esecutivo, come prevede la Costituzione. *(Applausi

Le chiedo, quindi, Presidente, di farsi portavoce con il presidente Marini e con il Consiglio di Presidenza perché anche il Senato possa essere dotato di questo strumento che permette di far conoscere il nostro lavoro

opportuni contatti e garantire la diretta televisiva. Mi mandi una richiesta e cercherò di dare un seguito